di presentazione PRESIDENTE. Comunico che in data 9 settembre 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri: «Conversione in legge del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»

quindi chiederei una proroga. Ci rivedremo alle 18,30 per lavorare in Commissione, andando avanti quanto possibile e necessario, nella misura in cui ciò si rivelerà proficuo.